per esprimere il nostro profondo cordoglio per la scomparsa, il 23 febbraio scorso, nel Policlinico San Matteo a Pavia, del professor Giovanni Ferrara. Egli è stato per tre legislature, a partire dal 1983, senatore della Repubblica per il Partito Repubblicano. Dal 1992 al 1994 mi fu vicino in questi banchi. apparteneva ad una notissima famiglia romana, laica e antifascista. Il padre Mario fu un eminente avvocato liberale, amico di Giovanni Amendola. Giovanni Ferrara ebbe due vocazioni dominanti: quella di studioso di storia antica, che gli procurò la prestigiosa cattedra in questa disciplina all'Università di Firenze, e quella di politico fermamente legato alla tradizione della democrazia repubblicana e liberale. Saggista acuto e rigoroso, fu collaboratore de «Il Mondo», de «L'Espresso» e del quotidiano «la Repubblica». Il suo libro più noto, «Apologia dell'uomo laico», è un notevole e attualissimo saggio di moderna cultura liberale. fu sempre al fianco di Ugo La Malfa, di Bruno Visentini e di Giovanni Spadolini nelle loro lunghe battaglie politiche. Ha ben scritto il presidente della Repubblica Napolitano: «La pacatezza e la serenità, che erano componenti essenziali del suo stile personale, si sono sempre coniugate con la coerenza e la fermezza delle idee e dei comportamenti». Si può dire che, fino all'ultimo, la sua passione lo ha portato ad impegnarsi senza risparmio. Il suo malore, infatti, è nato dopo una lezione alla Scuola di formazione politica di Libertà e Giustizia. Esprimo il nostro rimpianto per un uomo che ha onorato il nostro Parlamento e che nella politica italiana è stato un vivido esempio di coerenza e di rigore intellettuale e morale.

Colleghi, la Conferenza dei Capigruppo, riunitasi questa mattina, ha approvato all'unanimità modifiche ed integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino a giovedì 15 marzo. Oggi pomeriggio riprenderà la discussione del decreto-legge per la prevenzione della violenza nelle competizioni calcistiche. A conclusione del decreto-legge, nella giornata di domani saranno posti all'ordine del giorno i disegni di legge sul procedimento ingiuntivo, sulla modifica dell'articolo 27 della Costituzione per l'abolizione della pena di morte, nonché due ratifiche di accordi internazionali. Resta confermato che nella giornata di giovedì 8 marzo l'Assemblea non terrà seduta, su richiesta delle onorevoli senatrici. Le Commissioni potranno convocarsi a condizione dell'unanimità dei Gruppi in esse rappresentati e con l'assenso delle senatrici componenti. Per quanto riguarda i lavori della prossima settimana, nella seduta pomeridiana di martedì 13 marzo sarà discussa una proposta di risoluzione che la 14a Commissione permanente si accinge a votare sui principali temi dell'Agenda politica europea. In apertura della seduta antimeridiana di mercoledì 14 marzo, avrà luogo la votazione - mediante schede, col sistema delle urne aperte - per l'elezione di due senatori Segretari, ai sensi dell'articolo 5, commi 2-*bis* e 2-*ter*, del Regolamento. L'intera giornata sarà poi dedicata all'esame del decreto-legge sull'attuazione di obblighi comunitari e internazionali, per il quale si è proceduto alla ripartizione dei tempi tra i Gruppi. Ove non conclusa, la discussione proseguirà martedì 20 marzo. Nella seduta antimeridiana di giovedì 15 marzo saranno discusse mozioni in materia di politica ambientale. È stato infine stabilito che la votazione per l'elezione di quattro componenti effettivi e quattro supplenti della Commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti abbia luogo nella giornata di mercoledì 21 marzo, in concomitanza con l'analoga votazione della Camera dei deputati.

quanto accaduto in Afghanistan, anche alla luce di alcune dichiarazioni di esponenti della maggioranza, molto critiche nei confronti del Governo, ma lei mi ha preceduto. Aspettiamo

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo». «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo ad eccezione delle proposte 2.33, 2.37, 9.0.1 (limitatamente al comma 6), 9.0.2 (limitatamente al comma 3), 11.0.3 (limitatamente alle parole: "essere in possesso dell'attestato di qualifica rilasciato dal Comitato regionale di vigilanza agenzie di sicurezza, di seguito Corevas di cui al successivo art. 135" di cui al comma 2 del capoverso "art. 134", nonché ai capoversi "art. 135, 136 e 137") e 11.0.2 (limitatamente al capoverso "art. 11-*quater*", comma 1, lettera *d*) sulle quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nonché della proposta 1.12 sulla quale il parere è contrario. Sull'emendamento 11.0.2 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, a che nel capoverso "art 11-*bis*", dopo le parole: "il Ministro dell'Università e della ricerca e con il Ministro delle politiche per la famiglia predispone" siano inserite le parole: "senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"».

fosse quello di impedire che si formino dei pullman che vadano in altre città. Questo obiettivo viene garantito e salvaguardato,

a stabilire una situazione simile a quella degli stadi inglesi. È noto che in Inghilterra c'era il problema dei cosiddetti *hooligans*, che è stato in larga parte risolto adottando misure che intervengono a monte della repressione. In questo caso si ritiene inutile, ancorché controproducente, dividere i tifosi con delle barriere che, in alcuni casi, sono delle vere e proprie gabbie. Il nostro emendamento mira ad eliminare

Signor Presidente, ritiro l'emendamento 1.6 perché l'obiettivo che intendeva raggiungere è stato conseguito con l'emendamento 1.8 delle Commissioni riunite.

prevede dei requisiti per coloro che svolgeranno attività di sicurezza all'interno degli stadi, ma è anche vero che questi requisiti saranno definiti da un decreto del Ministro dell'interno che avrà dei tempi tecnici di elaborazione e, successivamente, è previsto un termine per applicarlo. Allora, sarei disponibile, se i relatori e il Governo concordano, a considerare l'emendamento 1.12, che aggancia i requisiti a quelli di chi ha la qualifica di guardia particolare giurata, per il periodo transitorio finché il nuovo regime non sarà pienamente operativo. Quello che non si può consentire, però, è che norme che sono immediatamente applicabili (da subito all'interno degli stadi sono chiamati ad operare i cosiddetti *steward*) non siano coperte da chiarezza sulla qualifica di chi deve svolgere questa funzione.

e presentiamo un provvedimento largamente condiviso. Il mandato che abbiamo avuto io e il collega Di Lello è un mandato unanime delle Commissioni riunite. È chiaro che gli emendamenti delle Commissioni riunite rappresentano un punto di mediazione politica che ha trovato la soddisfazione di tutti i Gruppi parlamentari.

richiesta un pochino curiosa, perché intanto non risponde a verità che vi sia stato un accordo unanime: c'è stato un accordo, che è stato corretto, larghissimo e ne prendo atto,

Signor Presidente, colleghi, nella tarda serata di ieri, la redazione del quotidiano "la Repubblica" ha comunicato all'unità di crisi della Farnesina di non essere riuscita a mettersi in contatto, da diverse ore, con il proprio corrispondente in Afghanistan, Daniele Mastrogiacomo. La testata ha specificato che Mastrogiacomo si era trasferito da Kabul a Kandahar per motivi di servizio. Appena ricevuta la segnalazione, sono partite immediatamente le ricerche, in stretta collaborazione con l'Ambasciata d'Italia a Kabul e i Servizi d'informazione. Nelle prime ore della mattina di oggi, «la Repubblica» ha precisato che i contatti con Mastrogiacomo risultano interrotti dalle ore 21 di domenica. Sono giunte da più parti, comprese fonti alleate, notizie che indicherebbero che due cittadini di nazionalità afghana, che potrebbero essere l'autista e l'interprete del giornalista italiano, e un occidentale di cittadinanza non specificata sarebbero stati trattenuti da un gruppo di talebani. Notizie di stampa avevano anche riportato, in un primo momento, come anche un cittadino britannico fosse stato sequestrato dai talebani: su quest'ultima notizia però vi è stata la smentita del *Foreign Office*. In questo momento la Farnesina, in stretto raccordo con le altre istituzioni interessate, sta attivando tutti i canali per accertare l'accaduto e rintracciare il Mastrogiacomo. I familiari sono stati, naturalmente, informati sia dalla redazione di «la Repubblica» che dall'unità di crisi. La questione è seguita personalmente e in tempo reale dal ministro degli affari esteri Massimo D'Alema. Alle ore 17,03 è stato diramato a Kabul un comunicato, attribuito al portavoce dei talebani Mohammed Yousuf, che parla di cattura di un giornalista italiano che lavora per «la Repubblica», con l'accusa, rivolta nei confronti del giornalista, di Sono in corso ovviamente anche su questo ultimo e recente comunicato, diffuso, peraltro, anche dalle agenzie in Italia, le necessarie valutazioni. Signor Presidente, colleghi, questo allo stato è quello che si può comunicare in maniera inequivoca all'Aula, fermo restando che, di minuto in minuto, alla luce alla luce degli approfondimenti, delle indagini, delle analisi, delle notizie e delle informazioni che arriveranno dall'Afghanistan, ci riserviamo di informare in tempo reale,

solo per aggiungere motivi di preoccupazione e di partecipazione a quanto riferito dal rappresentante del Governo, ma anche per ricordare un problema non è certo nuovo sui fronti di guerra sparsi in tutto il mondo: quello dell'assistenza e della tutela degli inviati dei giornali non solo italiani. di stampa confermano quanto ha detto testé il rappresentante del Governo ma in un'evoluzione tutt'altro che rassicurante per noi. Se, infatti, le prime fonti dicevano che era stato fermato un cittadino britannico, probabilmente giornalista, e con lui due afghani, forse un autista e un accompagnatore interprete, le ultimissime notizie di organi di stampa che provengono direttamente da Kabul parlano quasi certamente di un italiano

di essere delle spie pare sia stata ufficializzata. Questo chiaramente non può che turbarci profondamente, soprattutto in seguito agli avvenimenti che si sono susseguiti in queste ultime ore nella zona.

Anche un portavoce dei talebani, che negli ultimi avvenimenti è stato considerato degno di fiducia, Qari Yousof Ahmadi, fa l'ipotesi che il britannico sia proprio il giornalista italiano per il semplice fatto che ovviamente si esprime in inglese. Una conferma in questo senso è venuta anche dall'agenzia «France Press». Quello che ancora di più può essere motivo di turbamento è la recente mobilitazione dei cittadini dell'Afghanistan in seguito alle 21 vittime degli ultimi bombardamenti americani,

4.500 soldati NATO più 1.000 soldati afghani. Tutto questo non ha fatto che accendere dei sentimenti che non sono certo amichevoli nei confronti di chi partecipa a tali operazioni. Va ricordato che dall'inizio dell'anno in quella zona si sono registrate ben 21 vittime tra i soldati stranieri, non afghani.

al programma ambizioso dell'«operazione Achille» finalizzato a combattere il mondo della droga e la produzione dell'oppio, non favorisce la serenità per affrontare questo episodio che ci riguarda direttamente. La mobilitazione della popolazione, si sa, può infiammare gli animi e può anche motivare

Signor Presidente, intervengo per esprimere, a nome del Gruppo Per le Autonomie, la forte partecipazione e la solidarietà nei confronti del giornalista rapito, dei suoi familiari e dei colleghi giornalisti de "la Repubblica", insieme, naturalmente, alla grande preoccupazione per quanto sta accadendo in Afghanistan. Non credo però sia questo il momento di anticipare una discussione che svolgeremo in modo disteso nei prossimi giorni, sia nelle Commissioni esteri e difesa che in Aula, in occasione del dibattito sul rinnovo delle missioni italiane all'estero. Certamente è difficile non mettere in collegamento questo episodio con gli avvenimenti dei giorni scorsi, che rivelano un uso che potrebbe essere politicamente inavvertito della forza militare. È evidente che è impensabile stabilizzare la situazione irachena senza il ricorso ad una forza armata multilaterale ed internazionale; tuttavia è del tutto evidente anche che questa forza deve essere impiegata avendo sempre presenti gli obiettivi politici che ci si propone. Il principale obiettivo politico è quello di stabilire un'alleanza forte con le popolazioni, che isoli le componenti fondamentaliste e in particolare quella dei talebani in Afghanistan. Gli episodi cui abbiamo assistito nei giorni scorsi, invece, ci fanno balenare la preoccupazione che possa accadere il contrario, cioè che di fronte ad attacchi che non discriminano tra terroristi o insorgenti talebani e cittadini inermi vi possa essere una saldatura che va all'opposto. all'opposto. In questo momento, dobbiamo evitare di ragionare sulle misure politiche ed anche militari che dovremo assumere nei prossimi giorni, lasciandoci prendere dal ricatto che evidentemente questo rapimento comporta. Quindi, dobbiamo riuscire a mantenere la doverosa e necessaria serenità dal punto di vista politico e istituzionale, che in questo momento non può non associarsi all'impegno più forte in favore della liberazione del nostro concittadino

identificazione tra la funzione del giornalista e quella della spia, che è assolutamente inaccettabile e irricevibile. *(Applausi Signor Presidente, onorevoli colleghi, a nome del Gruppo Insieme con l'Unione esprimo la nostra solidarietà al giornalista Daniele Mastrogiacomo, alla sua famiglia e alla testata,

pedine più importanti sullo scacchiere dei conflitti. Non a caso abbiamo inventato quell'oscenità, deontologicamente insulsa, che si chiama il giornalista *embedded*; non a caso molti Governi hanno approntato agenzie di disinformazione

è che la non verità è un dato essenziale della guerra. Quindi, dovremo iniziare a riflettere seriamente su come poter garantire un minimo di informazione democratica, una pluralità delle fonti,

come ciò che è negato - l'informazione è tappa fondamentale di questo tempo di guerra e di dominio: poiché la verità - scusatemi - è sempre rivoluzionaria anche quando non ci piace, è davvero una delle vittime, insieme agli operatori di verità e di informazione,

vadano fatte, cercando di rispettare - almeno per quanto è possibile - l'oggettività delle cose. Intanto, ho sentito il vice ministro Danieli usare un termine pudico: sono stati «trattenuti». Vice ministro Danieli, sono stati rapiti! Credo che questo sia il dato fondamentale che dobbiamo considerare. Allora dobbiamo pensare in che modo in questo momento si sta evolvendo la situazione in Afghanistan. Si era detto che sarebbe partita la controffensiva talebana di primavera. Ebbene, questo è evidentemente un episodio che fa parte a tutti gli effetti di questa controffensiva.

Ho sentito dire da molte anime belle che in Afghanistan dobbiamo mandare più civili. Noi abbiamo messo in guardia avvertendo che i civili saranno indifesi se manderemo i nostri militari con le attuali

girano senza alcuna scorta, completamente indifesi. È del tutto evidente che la situazione si sta evolvendo verso una situazione di tipo iracheno, dove invece i civili venivano sempre e costantemente scortati dai nostri soldati. Questo è un dato. Non possiamo pensare che i nostri soldati stiano in Afghanistan come avete pensato voi per salvare la coscienza della sinistra radicale. Dobbiamo poter pensare che stiano in Afghanistan per compiere un servizio oggettivo e positivo, soprattutto per i nostri civili, altrimenti vi sarà una situazione paradossale per la quale i militari staranno chiusi nelle caserme e i civili in giro, senza difesa. difesa. Noi non potremo mai votare per una situazione di questo tipo e credo che la maggioranza, che ha la responsabilità politica di licenziare questo provvedimento, debba porsi tale problema. Non voglio usare parole forti, ma attenzione che il sangue dei civili che potrebbe essere versato - spero di no - in Afghanistan nei prossimi mesi potrebbe ricadere su quest'Aula se voteremo dei provvedimenti ipocriti!

Signor Presidente, sono opportune le comunicazioni del Governo su questo episodio di sequestro da parte dei talebani del giornalista Daniele Mastrogiacomo. Ancor più opportune tutte le iniziative che il Governo dovrà assumere e gestire per tentare di riportare Mastrogiacomo alla sua personale libertà e quindi alla possibilità di esercitare la sua funzione di giornalista e di informatore in termini pieni e completi. Ritengo inopportuno invece anticipare o condizionare il dibattito già aperto in Parlamento, in questo momento alla Camera dei deputati, sul rifinanziamento della missione in Afghanistan. Perché inopportuno? Perché è necessario, innanzi tutto (l'ho sentito dal senatore Tonini, lo apprezzo e lo condivido), evitare che l'episodio possa condizionare la libertà del Parlamento italiano. Conosciamo la missione in Afghanistan e le caratteristiche che essa ha avuto; il Parlamento dovrà stabilire in quale misura esse dovranno essere confermate e in quale misura potranno essere modificate, lo dico subito: difficilmente si potrà andare nella direzione di una pura missione di Croce Rossa, perché l'impegno che l'Italia ha assunto va gestito in continuità, ma va gestito anche con estrema capacità di adeguamento ad una situazione che, come tutti sanno, è in via di evoluzione. Da tempo, infatti, sappiamo che con la primavera ci sarebbe stata un'offensiva dei talebani; è probabile che questo episodio di sequestro sia anticipatore della strategia guerrigliera dei talebani. Evitiamo che esso condizioni la libertà con cui il Parlamento si deve muovere. Evitiamo però che questo episodio venga a consolidarsi e quindi ogni iniziativa, non soltanto del Governo italiano, ma del Governo italiano in rapporto alla NATO

a disegni - anche necessitati - unilaterali, che potrebbero portare anche alla ripetizione di episodi non del tutto felici e non del tutto positivi. È un momento in cui il Governo, il Parlamento e il Paese sono chiamati a un atto di grande serietà e di grande compostezza. È questa serietà e compostezza che determinano la solidarietà

la preoccupazione per la possibile controffensiva talebana, la preoccupazione per la sua incolumità fisica e per i rischi che correrà il nostro contingente presente ancora in Afghanistan (perché è evidente che la situazione andrà deteriorandosi anche a Herat e a Kabul, come ci dicono molte fonti dei Servizi segreti spagnoli e altro), la preoccupazione perché con l'avanzare della macchina della guerra della NATO si riducono al minimo le già minime possibilità di una soluzione negoziale e diplomatica al conflitto, della quale giustamente il nostro Paese oggi si fa portatore. La notizia del rapimento di Daniele Mastrogiacomo dimostra che l'informazione, come è stato detto molto chiaramente dal collega Silvestri, è una delle principali vittime collaterali della guerra. Lo avevamo sperimentato con il rapimento di Giuliana Sgrena in Iraq. Lo stiamo constatando alla luce della recente strage di civili ad opera di truppe statunitensi a Jalalabad, quando i *marines* hanno voluto cancellare con la forza le prove di quell'eccidio compiuto contro popolazioni civili inermi. Osserviamo impotenti lo sviluppo di un conflitto che probabilmente incendierà tutto l'Afghanistan. Rischiamo di dover sentire ancora notizie di danni collaterali, scuse ipocrite da parte dei portavoce ISAF e dovremo constatare che alla fine il popolo afghano, che in molti volevano andare ad aiutare, ci si ritorcerà contro, giacché quelle truppe sono sotto comando unificato americano e l'operazione «*Enduring Freedom*», che è parte dell'offensiva militare in Afghanistan, è sotto lo stesso comando del contingente ISAF, nel quale ci sono anche soldati italiani, che rischiano di essere visti anche loro come truppe di occupazione da parte della popolazione civile afghana. Avremo occasione di discutere a fondo in Senato nelle prossime settimane; discuteremo e proporremo modalità per trasformare la presenza internazionale in Afghanistan, un Paese ed un popolo che non vogliamo lasciare a se stesso, ma che vogliamo sia artefice del proprio destino e che possa vivere in sicurezza, pace e giustizia. Sosterremo l'iniziativa del Governo italiano per il rilancio della cooperazione civile, non soltanto con funzionari civili (la cooperazione civile si fa anche appoggiando la ricostruzione da parte delle stesse comunità afghane), e della diplomazia internazionale. Proprio perché in questo profondamente crediamo, oggi non possiamo non interrogarci sul rischio che la nostra presenza in Afghanistan, in quelle condizioni di guerra, dentro il contingente ISAF, sotto comando americano, possa diventare un ostacolo e non uno strumento verso quel fine di soluzione diplomatica, politica e civile del conflitto afghano sul quale noi vogliamo invece investire ancora di più. Di questo discuteremo, avremo tempo per farlo. Oggi rivolgiamo veramente un invito al Governo a fare tutto quello che è possibile per restituire Daniele Mastrogiacomo ai suoi colleghi e alla sua famiglia e per garantire la sua incolumità e che, anche in quel terreno di guerra, sia fatta verità e sia fatta luce. Invitiamo quindi il Governo ad essere pronto a continuare a venire a riferire in Parlamento in merito alle condizioni effettive che i nostri soldati oggi vivono in quel Paese.

perché dovremmo almeno sapere se Mastrogiacomo aveva concordato con il nostro contingente e con la Farnesina il suo spostamento, se era libero di muoversi senza nessuna scorta, se e perché i nostri soldati restano chiusi dentro le mura di una caserma e invece i civili possono tranquillamente girare, con i rischi conseguenti in un Paese pericoloso come l'Afghanistan. Ci consenta di esprimere tutta la nostra rabbia e anche il nostro fastidio per le posizioni radicali qui esposte, del tutto improprie, perché abbiamo letto delle agenzie che riportano la preoccupazione per l'offensiva USA, attacchi ai *marines* che fanno emergere più che mai l'anima antiamericana di questa parte della maggioranza, che è arrivata addirittura a proporre di di acquistare l'oppio, sapendo bene che alla fine non sarebbe altro che un finanziamento surrettizio ad Al Qaeda o ai talebani. Allora, noi vorremmo sapere, risentendo un'altra volta il ministro degli esteri Massimo D'Alema, cosa ne pensa della conferenza di pace, a questo livello con chi pensa di farla, con chi pensa di trattare, quando, come, e se se non ritenga che siano posizioni giusto per sollevare un po' di cortina fumogena, per cercare di tranquillizzare parte della propria maggioranza in vista di un voto che mostrerà la discontinuità e le divisioni di questa maggioranza. Oggi, non uno qualsiasi dei parlamentari e senatori di quest'Aula, ma il capogruppo di Rifondazione Comunista, il senatore Russo Spena, ci dice addirittura che il Governo dovrà spiegare, come non ha fatto finora, cosa fanno i nostri soldati lì, quali sono concretamente le attività di aiuto alla popolazione, qual è materialmente l'attività del contingente italiano. Queste iniziative sono concordate e trovano l'assenso anche di tante altre parti della maggioranza di questo Governo, che addirittura, come abbiamo sentito adesso dall'intervento del collega Martone, propongono nient'altro

Noi dobbiamo ribadire, ancora una volta, che la politica estera è il collante di una maggioranza: non ci può essere una maggioranza variabile in politica estera. Le maggioranze variabili possono esserci su problemi contingenti, su problemi quotidiani, su problemi tecnici; non ci possono essere su problemi che riguardano il ruolo dell'Italia, il diritto dell'Italia, le responsabilità che il nostro Paese si deve assumere davanti al mondo. Quindi noi, al di là di di esprimere ancora una volta la solidarietà e la preoccupazione nei confronti di questo bravo e valoroso giornalista, non possiamo far altro che ribadire la nostra preoccupazione per un Governo e una maggioranza che in politica estera sono totalmente allo sbando e mettono a repentaglio, anche con questo questo loro modo di fare e agire, la vita e l'incolumità dei nostri concittadini. Signor Presidente, anch'io, a nome del Gruppo di Forza Italia, voglio esprimere la mia solidarietà a Daniele Mastrogiacomo e comprendere anche l'apprensione e la trepidazione dei familiari per quanto sta accadendo al giornalista. Voglio altresì esprimere solidarietà ai giornalisti per il loro impegno per l'informazione. Capisco la delicatezza e la riservatezza con cui bisogna affrontare questo episodio e quindi non mi esimo dal senso di responsabilità nel fare questa valutazione, però

ci sono tante agenzie che hanno dato maggiori informazioni. Tra l'altro c'è da dire che il giornalista aveva raccontato nei giorni scorsi quale era il suo possibile impegno come giornalista in quell'area così delicata.

in ragione del fatto che, come sappiamo benissimo e anche la stessa procura della Repubblica ha immaginato, se il sequestro - riferiva poc'anzi un'agenzia venisse confermato (e ormai mi pare che sia confermato), si tratterebbe di un sequestro di persona con finalità di terrorismo.

oltre ad una tempestività di informazione, anche maggiori ragguagli. Sappiamo che in questo momento c'è la necessità

abbiamo appreso del rapimento di Daniele Mastrogiacomo con angoscia ed emozione, sentimenti che in queste ore saranno certamente forti nella sua famiglia, nella redazione di «la Repubblica», nel Paese, che ha già vissuto momenti del genere, - se permettete - anche in quelli, tra noi parlamentari, che ne condividono la professione o - come nel mio caso - sono stati suoi compagni di lavoro nella stessa redazione per tanti anni e ne conoscono la serietà, l'impegno e la libertà.

tentava (come leggevamo su «la Repubblica») di mettere in luce il punto di vista degli afghani, delle popolazioni di quel Paese. Il rapimento, e il modo protervo con cui è stato annunciato e rivendicato, conferma a tutti noi che in Afghanistan l'obiettivo primario, fissato dalle Nazioni Unite e affidato alla NATO, quello di garantire la sicurezza nel Paese, è ben lungi dall'essere raggiunto. A mio modo di vedere, questa è un'ottima ragione per moltiplicare i nostri sforzi in questa direzione, sia dal punto di vista militare (perché non c'è altro modo di fermare un uomo in armi che un altro uomo in armi), sia dal punto di vista politico e civile. Infatti, la comunità internazionale ha fatto scandalosamente poco per la ricostruzione dell'Afghanistan in questi anni: in tutto il mondo, abbiamo speso 57 dollari *pro capite* all'anno per ricostruire l'Afghanistan.

fino in fondo quale dovere morale il mondo democratico abbia nei confronti del popolo afghano: esso non può essere lasciato in balia della guerra civile e dell'obbrobrio del regime talebano per la seconda volta nella sua storia dopo la cacciata dei sovietici. Al tempo stesso, bisogna avviare una strategia nuova - questa sì, nuova - per la conquista dei cuori e delle menti degli afghani, cioè di quella ampia area grigia del Paese che certo non sta con i talebani, ma che oggi non sta nemmeno con la coalizione internazionale.

Come in altre occasioni, dobbiamo mostrare che il Parlamento e la politica non sono l'anello debole del sistema Paese italiano. Abbiamo il dovere di dare assoluta priorità all'interesse nazionale della protezione della vita e della sicurezza dei nostri connazionali in Afghanistan e alla liberazione di Daniele Mastrogiacomo. Tutto il resto viene dopo, a mio modo di vedere. Sono certo che il Parlamento saprà farlo anche questa volta. una nuova finestra"). Il Senato, colleghe e colleghi, mi pare abbia espresso nel modo più solenne e unanime la preoccupazione per quanto sta avvenendo, ovviamente la Presidenza fa proprio l'invito al Governo a seguire con continuità la vicenda e a trovare le strade, se è possibile (noi ci auguriamo che lo sia), per salvare, intanto, la vita del giornalista e permettere che continui la propria importante attività.

Signor Presidente, poiché è stata interrotta la procedura ordinaria, nel senso che essendo mancato il numero legale noi avremmo dovuto riprendere dopo venti minuti ma la Presidenza ha deciso di far svolgere questa giusta e doverosa comunicazione al Governo, con gli interventi che sono soltanto se potesse dare un avviso che si riprende con la procedura ordinaria e con immediate votazioni, in maniera che i colleghi che sono in giro per il palazzo

Presidente, raccomando l'approvazione di questo emendamento. Trovo contraddittorio il parere contrario del relatore: infatti egli dice compete agli *steward* la sicurezza interna agli stadi (e su questo siamo tutti d'accordo), ma il problema è che oggi gli *steward* preparati non sono disponibili, e un altro emendamento, il 2.0.500, approvato già in Commissione, si demanda ad un decreto di indicare le loro qualità soggettive. L'emendamento 1.12 punta a colmare il regime transitorio, non a trasformare gli *steward* in guardie particolari giurate. Vorrei capire cosa succede nel periodo intermedio, quando non c'è la qualificazione, non c'è la preparazione e c'è il rischio che squadre di tifosi organizzati vengano incaricate dalle società sportive di svolgere questo ruolo. PRESIDENTE. Il relatore ha qualcosa da aggiungere? Presidente, non posso che ribadire quanto ho già detto alle Commissioni riunite. Noi abbiamo fatto un accordo unanime intorno all'emendamento 2.0.500 delle Commissione riunite e abbiamo deciso tutti insieme di differire la questione degli *steward* ad un decreto del Governo per il quale abbiamo chiesto di dare il parere alle Commissioni competenti di Camera e Senato. I colleghi hanno ritenuto, me compreso, che non fosse utile si qualificasse come guardia giurata colui che sta all'interno degli stadi al posto della polizia: non ci sembrava utile e non ci sembra nemmeno necessario, anche perché nel regime transitorio c'è il decreto‑legge che prevede si applichi l'articolo 11 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e ci sono i decreti attuativi del decreto-legge Pisanu, quindi la disciplina che si è applicata in questa materia nelle settimane precedenti. Reputo pertanto totalmente destituito di fondamento

di applicare la misura del divieto di accesso agli stadi, prevedendosi che la stessa cosa possa essere disposta anche in assenza di denuncia o sentenza di condanna. Tale disposizione va a novellare l'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, nella parte in cui subordina l'applicazione della misura *de quo* all'esistenza di una denuncia o condanna: infatti, nella novella prevista dalla norma che abbiamo di fronte, è possibile arrivare allo stesso risultato sulla base di elementi oggettivi diversi dalla denuncia o dalla condanna. Però la fattispecie che ci occupa e della quale io, come i colleghi di Rifondazione Comunista, chiedo l'abrogazione, resta comunque una misura interdittiva disposta per la salvaguardia di finalità inerenti all'ordine pubblico. Tale indiscussa natura non rende opportuno prescindere, ai fini applicativi, quantomeno dall'esistenza di una denuncia per specifici reati. Giova sul punto evidenziare - ma non sarà sfuggito assolutamente alla Commissione e ai relatori - che il codice di rito, per il tramite dell'articolo 280, subordina ancora l'applicabilità delle misure coercitive all'apertura di un procedimento penale per delitto punito con la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni; nel caso di specie, invece, questa misura verrebbe applicata, come detto, sulla base di elementi oggettivi molto particolari ed indefiniti. Riteniamo che una norma come questa - e mi rivolgo chiaramente ai relatori - potrebbe tranquillamente essere espunta dal provvedimento, perché non mi pare che sia quella che lo caratterizzi in maniera decisiva.

illustro, in via del tutto generale, una serie di proposte che sono diversamente formulate per poter dare all'Aula la possibilità di valutarle e di votare quella ritenuta più equilibrata. Sostanzialmente gli emendamenti intervengono su un tema che io ritengo assolutamente delicato, sia per la sostanza sia perché si è dimostrato, ad esempio negli stadi inglesi, quello decisivo per il buon andamento delle partite: mi riferisco ai cosiddetti assistenti, o *steward*, o come li vogliamo chiamare. È chiaro che questi incaricati svolgono un compito delicatissimo: pensiamo soltanto al fatto che hanno la facoltà di intervenire in qualche modo sui tifosi intemperanti con tutto quello che ne consegue e anche con i rischi a cui sono sottoposti, perché è già accaduto che alcuni volontari, in occasioni peraltro diverse (penso per esempio ai volontari bolognesi che, tra l'altro, stati istituiti dal sindaco Cofferati), per il semplice fatto di aver contribuito all'ordine pubblico si sono trovati incriminati dalla magistratura. Allora è ovvio che questi incaricati devono avere una solida preparazione professionale, devono sapere esattamente quello che devono fare e avere un notevole sangue freddo, perché agiscono in condizioni

e proponiamo anche che, in prima battuta, tale compito possa essere svolto da chi già svolge funzione di vigilanza. A questo proposito, francamente ci siamo stupiti del fatto che sia il relatore sia la Commissione non abbiano inteso addivenire a questa soluzione perché sicuramente chi già svolge compiti di vigilanza ha una solida preparazione professionale proprio in tal senso. Per questo sollecitiamo l'Assemblea ad approvare soprattutto l'emendamento che prevede anche l'impiego di addetti agli organi di vigilanza in queste fattispecie. Presidente, tutti gli emendamenti all'articolo 2 presentati a mia firma sono da considerare ritirati perché in Commissione sostanzialmente

aggravare le sanzioni a carico di chi commette fatti gravi durante lo svolgimento di gare; punire le società che concorrono a tenere rapporti con associazioni di facinorosi. La linea di fondo è distinguere i tifosi dai facinorosi.

alla luce delle spiegazioni che lì erano state fornite. Abbiamo chiarito che si intende incidere sulle facoltà e non sulle libertà e sui diritti; infatti non stiamo parlando di vietare i i diritti fondamentali delle persone, ma stiamo vietando a persone che hanno commesso delle violenze all'interno degli stadi di tornarvi, ancorché abbiano ricevuto una denuncia e non una sentenza passata in giudicato. Se si trattasse di una libertà, converrei con le argomentazioni

quella è l'occasione in cui, con i colleghi di maggioranza e opposizione, abbiamo convenuto di aprire un confronto e discutere di cosa dovranno fare gli *steward*.

Presidente: non ritiro questo emendamento perché, in questo momento, stiamo parlando del divieto di partecipazione alle manifestazioni sportive, che dalla giurisprudenza, anche di legittimità, viene qualificato come una misura di prevenzione.

perché si parla di «chi, sulla base di elementi oggettivi, risulta avere tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive». Non è la descrizione di un reato, altrimenti ci troveremmo di fronte a qualcosa che ha una sanzione penale, e non è la descrizione di un tentativo di reato, perché contiene soltanto una parte di un tentativo di reato; manca la direzione univoca di questi atti. Il testo che mi permetto di proporre all'Aula è più conforme

sicurezza interna di impianti sportivi all'articolo 11 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Ora, questo articolo prevede il diniego al rilascio di autorizzazioni - e in questo caso si fa riferimento ai requisiti che consentono il rilascio di autorizzazioni a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto doloso e a chi è sottoposto all'ammonizione (che non esiste più) o a misure di sicurezza personale, o sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza. Se vale il riferimento a questa norma, chi ha patteggiato per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa può fare l'addetto alla sicurezza interna agli stadi perché, avendo le attenuanti o anche, senza necessità di attenuanti, la diminuente di pena prevista per il minimo edittale dell'associazione mafiosa, si è al di sotto del limite dei tre anni di reclusione. Le altre ragioni ostative, cioè la dichiarazione di delinquente abituale, professionale o per tendenza sono qualifiche molto impegnative che richiedono la consumazione di reati abbastanza gravi. Con l'emendamento 2.22 si propone semplicemente il rinvio agli elementi che consentono il rilascio della qualifica di guardia particolare giurata.

un'intesa in Commissione in base alla quale le questioni relative alla violenza nei confronti delle cose sarebbero state trasformate in un'aggravante del delitto di danneggiamento.

la norma punisce chiunque lancia o utilizza negli impianti sportivi o nelle immediate adiacenze razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi e così via.

qualcuno lancia un bengala all'interno di uno stadio con migliaia di spettatori, il pericolo è insito in questa condotta. Da ciò nasce l'emendamento 3.1, che propone di sopprimere questo inciso.

per i fatti previsti. Sappiamo tutti, però, che nessuno sarà mai condannato all'effettiva reclusione e quindi questa diventa la solita grida manzoniana. Abbiamo proposto, pertanto, di aggiungere una sanzione pecuniaria, che a a discrezione del giudice possa essere comminata. Credo sarebbe un deterrente molto più efficace della pura e semplice reclusione che, come sappiamo tutti, non viene mai applicata.

Presidente, con l'emendamento sottoposto all'Assemblea si vuole evidenziare il pericolo che l'arresto in flagranza venga consentito anche nell'ipotesi delittuosa di possesso di materiale pirotecnico. La vecchia norma di cui all'articolo 8 consentiva l'arresto nelle sole ipotesi di lancio di materiale pericoloso,

giudiziaria la facoltà di arrestare chiunque venga colto in flagranza di reato soltanto nelle ipotesi di reato con una pena della reclusione superiore al massimo a tre anni. Nella fattispecie, anche come modificata dalla normativa che stiamo esaminando, esaminando, il previsto aumento di pena da sei mesi a tre anni non sembrerebbe comunque astrattamente sufficiente a rendere possibile l'applicazione della misura, cioè a superare la preclusione di cui all'articolo 381 del codice di procedura penale. Anche questa sollecitazione viene fatta alla Commissione, fermo restando che il presentatore degli emendamenti non vuole mettersi in conflitto con le Commissioni riunite o con i relatori; ha soltanto la necessità di evidenziare una serie di problematicità

tale emendamento, nella percezione del fatto che i danni interni allo stadio possono riguardare non solo le persone, come tutto il provvedimento prevede, ma anche le cose.

Da questo punto di vista, si tratta di un'aggravante molto importante che cerca di sottolineare come anche la violenza nei confronti delle cose destinate allo svolgimento delle gare faccia parte delle sanzioni

è fastidioso, oltre che con gli sms, anche di persona! PRESIDENTE. Non mi costringa a censurarla, senatore Manzione. Il collega Boccia non è fastidioso ed è estremamente piacevole e collaborativo. si prevede, in relazione al reato di ingresso e permanenza negli impianti sportivi in violazione del relativo regolamento d'uso, la possibilità di applicare le misure del divieto di accesso e dell'obbligo di presentazione alla L'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, imponendo alla persona che vi è sottoposta un comportamento positivo, va sicuramente a limitare direttamente la libertà personale, seppure in modo meno invasivo delle misure detentive: dalla limitazione della libertà personale discende la necessaria applicazione di garanzie previste dall'articolo 13 della Costituzione. Ecco perché è stato presentato questo emendamento abrogativo che, ancora una volta, si rappresenta alle Commissioni riunite che, sappiamo, hanno lavorato benissimo per evidenziare una perplessità che non vorremmo un domani

Invito ancora il senatore Manzione a ritirare il suo emendamento. Si tratta in buona sostanza di consentire che si abbia uno strumento che si applica anche al di fuori delle celebrazioni delle manifestazioni sportive. La violazione del regolamento d'uso si può applicare anche quando lo stadio non è aperto, ma quando è chiuso. È evidente che può servire proprio ad impedire che si costituiscano le condizioni per commettere successivamente delle violenze. delle violenze. Le Commissioni hanno discusso se il divieto di andare allo stadio sia in realtà una violazione delle libertà personali o una mera violazione delle libertà di circolazione, tutelate non dall'articolo 13, ma dall'articolo 16 della Costituzione. Noi abbiamo preferito mantenere, anche alla luce di una giurisprudenza costante della Corte costituzionale - che non ha mai messo in discussione la validità di questo istituto - di confermare tale orientamento e di consentire che sia applicato anche in queste circostanze. Esprimo parere favorevole

capacità di inquadrare le fattispecie all'interno di una logica di princìpi. Ne prendo atto. C'è una volontà quasi unanime, non mi sento di insistere più di così.

l'emendamento 6.100 si evidenzia il paradosso di prevedere l'applicazione della misura di prevenzione nei confronti di chi agevola le condotte violente, non anche di chi le pone in essere.

obiettivamente c'è un'improprietà di riferimento per quanto riguarda il provvedimento di confisca. Anche in questo caso ci sembra un uso improprio di uno strumento che nasce con modalità assolutamente diverse. Rappresento all'Aula queste due esigenze. Capisco la necessità di licenziare al più presto il provvedimento e ne prendo atto, l'importante è che tali emendamenti restino agli atti.

Presidente, ringrazio la collega Boccia per le sue osservazioni. Abbiamo discusso a lungo dell'articolo 6. In Commissione abbiamo dato un'apertura di credito alle osservazioni che sono state formulate, e cioè che si tratta di una misura che si può applicare residualmente anche a quei soggetti che per un verso sfuggono al divieto del DASPO e per altro verso al reato che appunto consentirebbe l'arresto. In questi termini e tenendo presente che ci sono organizzazioni di ultras che comunque si configurano come organizzazioni di tipo criminale, invito il collega Manzione a ritirare i suoi emendamenti per favorire il mantenimento del testo presentato dal Governo.

ad aumentare notevolmente le sanzioni penali a carico di chi provocasse lesioni alle forze dell'ordine e che si è ritenuto di ricomprendere nell'ambito della norma generale, prevedendo un incremento di sanzioni. Ho dichiarato che ero soddisfatto perché il principio era stato colto e da questo punto di vista l'emendamento 7.8 può essere considerato ritirato, perché vi è una norma prevista dalla Commissione che consente di affrontare il problema in modo più che sufficiente.

del risultato raggiunto con l'inasprimento delle pene per chi procuri lesioni a pubblico ufficiale. Questo era l'obiettivo che ci eravamo proposti; quindi è stato raggiunto un grande risultato, dopo le vicende tragiche di Calabria e Catania.

Presidente, mi riservo di motivare il voto all'emendamento 7.6; preciso però da subito che, rispetto all'articolo 341 del codice penale che si ripropone,

Chiunque procuri ad un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico lesioni personali gravi o gravissime». Prendo atto del fatto che sono stati ritirati i successivi emendamenti. Credo di dover dare un parere soltanto sull'emendamento 7.6

sostanzialmente prevede che l'offesa possa essere arrecata e costituire oltraggio, quindi perseguibile d'ufficio e non a querela, soltanto quando le forze dell'ordine sono in servizio di ordine pubblico. Abbiamo creduto in Commissione che questo creerebbe una grave disparità di trattamento; mi rifaccio a quanto si diceva una volta: il bene giuridico tutelato non può essere la mansione, ma la funzione. Mi auguro che l'emendamento possa essere ritirato e trasformato in un ordine del giorno. Invito il Governo a rivalutare positivamente la possibilità di introdurre norme di tutela rafforzate nei confronti dei tutori dell'ordine, ma in un contesto tecnicamente più corretto e in una sede diversa da quella in cui stiamo discutendo quest'oggi. Mi auguro che il mio invito possa essere accolto

che non mi risulta essere strumento giuridico che possa avere la stessa efficacia di una norma penale. Non ho mai visto una sanzione applicata in virtù di un ordine del giorno, neanche nei confronti dei destinatari dell'ordine del giorno. Questo emendamento punta a reintrodurre nel nostro ordinamento, ma in modo molto più circoscritto, il reato di oltraggio a pubblico ufficiale che improvvidamente ne fu espulso qualche anno fa. Il testo che viene proposto all'Aula non è la fotocopia di quel testo abrogato, ma è una previsione molto più circoscritta - come ricordava il relatore - a quella esposizione esterna dei tutori dell'ordine in attività particolarmente rischiose. Non riguarda, quindi, per intenderci, il vigile urbano che eleva la contravvenzione per divieto di sosta. Trovo incongrua incongrua la motivazione del relatore secondo cui non si può limitare l'applicazione di questa norma alle funzioni di ordine e di sicurezza pubblica, quando abbiamo appena approvato un emendamento delle Commissioni riunite che prevede una fattispecie applicabile a chiunque procuri a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico lesioni gravi o gravissime. La previsione è assolutamente sovrapponibile e punta a introdurre un'ipotesi intermedia, prima di aspettare che l'autorità giudiziaria intervenga quando il pubblico ufficiale viene trattato con la spranga. Qui si sta individuando l'ipotesi in cui il pubblico ufficiale è destinatario di ingiurie, di sputi, di tutti quegli atteggiamenti che sono lesivi non soltanto della sua personale dignità, ma anche della dignità della divisa che indossa e di ciò che essa rappresenta. rappresenta. È assolutamente coerente con emendamenti già approvati, da ultimo il 7.200 (testo 2). Trovo singolare che il Governo in Commissione su questo emendamento si sia rimesso al Senato e in Aula manifesti invece la sua contrarietà aderendo al parere espresso dal relatore. In Commissione si è anche sentita la motivazione contraria da parte dei relatori (che per fortuna non è stata ripetuta in quest'Aula), secondo cui le organizzazioni sindacali non l'avrebbero richiesto, come se sottolineare un'esigenza sia necessaria la sollecitazione delle organizzazioni sindacali, che comunque si sono espresse e hanno chiesto a gran voce l'introduzione di questa norma. Non vorrei, ma ho il il leggero e fondato sospetto che questa sia la ragione principale per cui l'opposizione è contraria, non nel merito, ma in virtù di quell'ipoteca ideologica che grava su tutte le questioni di ordine pubblico e di sicurezza dall'avvio della legislatura a causa della consistente presenza in quest'Aula della sinistra estrema. Per questa ragione sollecito, nell'interesse delle Forze di polizia e della sicurezza della Nazione, il voto a favore di questo emendamento.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho trovato molto convincenti e motivate le considerazioni che ha fatto poco fa il collega, quale ha voluto sottolineare una posizione che non attiene ad una mansione (come ho sentito dire con una certa approssimazione dal relatore), ma all'effettività di una funzione nella fase più delicata e importante che vi possa essere, quella cioè di frapporre la dignità e la funzione dello Stato alle aggressioni fisiche, verbali, oltraggiose, che hanno un significato particolare in determinate condizioni e situazioni. Io sono stato tra coloro che hanno ritenuto che il vecchio reato di oltraggio avesse una motivazione, questa sì, qualche volta ideologica: della Polizia che debba fare più paura che incutere rispetto. Ma quando la funzione della Polizia è quella di garantire l'ordine democratico all'interno di una situazione così difficile e difficilmente controllabile, nella realtà di una folla in tumulto, di una situazione grave, non gratificare - mi permetto di dire - questa funzione con una valutazione di tutela, di garanzia, mi sembra una cosa abbastanza grave. Non sono d'accordo con il collega Mantovano nel ritenere che in quest'Aula ci debba essere una una situazione del tutto ideologica. Non credo che su materie giuridiche vi debbano essere bardature ideologiche. È un problema che riguarda un'attività di lavoratori della Polizia (mi permetto di usare questo termine).

perché si può aver avuto nella nostra storia, nella nostra visione filosofica della vita e della società, un'interpretazione che può essere stata anche giusta in certi momenti, quando la Polizia poteva rappresentare qualcosa di oppressivo, invece che di garanzia democratica. Per questo, credo che quest'emendamento debba essere accolto.

Io ho chiesto ai colleghi in Commissione di favorire le condizioni per l'immediata approvazione di questo decreto e di non introdurre argomenti nuovi o diversi da quelli trattati o presentati. Alla luce di questo, ho invitato a ritirare

Fatta questa premessa, signor Presidente, l'emendamento è anche tecnicamente sbagliato e lo dico al senatore Biondi, che ha ritenuto di dovervi aderire. Infatti, come ho detto, non è corretto tutelare la mansione e non la funzione.

fa l'operatore in servizio di ordine pubblico e chi, eseguendo una perquisizione a casa di un mafioso e ricevendo lo stesso oltraggio, è invece perseguito a querela e non d'ufficio. Con riferimento a questa ingiustizia,

vanno tutelati in quanto servitori dello Stato. In relazione a tale esigenza ho chiesto di fare un approfondimento in altra sede, rafforzando questa richiesta anche attraverso un invito al Governo. Questo intendimento era soprattutto

delicata e, in un contesto come questo, abbiamo esaminato questo decreto-legge alla luce di due considerazioni di fondo. Non si è trattato di un decreto-legge totalmente nuovo rispetto all'intervento promosso dal collega Pisanu quando era ministro dell'interno, perché sostanzialmente vi è un'importantissima continuità di reazione alla violenza negli negli stadi o nei dintorni degli stadi, e abbiamo voluto evitare fino in fondo che si creassero contrapposizioni all'interno delle due Commissioni, che pure hanno segnato gran parte della storia di questo Paese.

dal punto di vista normativo, uno strumento di pari efficacia rispetto ad un emendamento, ma noi stiamo per varare un decreto-legge che contiene numerose e significative norme di potenziamento dell'attività delle forze dell'ordine nel contesto delle manifestazioni sportive, quindi non si tratta di un ordine del giorno per non affrontare il problema, ma per affrontare il problema in termini diversi. Vorrei che questo punto fosse colto: non si tratta di ripristinare parzialmente l'oltraggio a pubblico ufficiale soltanto nell'esercizio delle funzioni, come è qui scritto; si tratta di un istituto che è stato abrogato nel 1999, la cui abrogazione ritengo parte di una cultura del lassismo che ha caratterizzato la vita politica italiana per molti anni e in questo momento mi sembrerebbe improprio pretendere di reintrodurre legislativamente una norma cancellata pochi anni fa, ma è molto importante dal punto di vista politico che ci sia un ordine del giorno condiviso dalla stragrande maggioranza dei senatori (probabilmente da tutti) che inviti il Governo seriamente a ripensare questa questione, non soltanto nell'esercizio delle funzioni, ma generalmente in quanto tutori dell'ordine pubblico. Lo dico perché mi sembra che questo sia il modo migliore per aiutare il Paese a uscire da una drammatica spirale di contrapposizione sulle forze dell'ordine, spirale dalla quale stiamo uscendo da qualche tempo, perché noto con piacere che man mano che vi è un richiamo ai nostri militari impegnati all'estero e alle forze dell'ordine, vi è in quest'Aula un notevole consenso che si va espandendo, a differenza di molti anni fa, quando su questo tema ci si divideva. Se vogliamo perseguire la linea di una intesa sulla tutela delle forze dell'ordine è meglio oggi fare il piccolo passo dell'ordine del giorno, anziché vedere bocciato un emendamento nella logica della contrapposizione. Questa è la ragione per la quale chiederei al relatore Sinisi di dire se l'ordine del giorno possa, come io ritengo, contenere espressamente la previsione anche di un ripristino alla luce di considerazioni generali, perché questo è un compito che si dà al Governo sapendo che ha alle spalle un voto molto largo dell'intero Senato. *(Applausi del senatore Eufemi).* non avrei preso la parola nel merito, perché mi ritrovo esattamente nelle considerazioni che ha fatto il mio collega di Gruppo, il senatore senatore Biondi. Vorrei però dire che nel metodo - e a volte le parole sono pietre - mi sembra che alcune affermazioni del relatore siano quantomeno eccessive. Sono uno che considera tutto il peso dall'appartenenza a un Gruppo partitico. Così come il vecchio Gladstone, credo che un gentiluomo, tra la propria coscienza ed il proprio partito, debba scegliere il proprio partito, ma non dimentichiamo che l'esercizio del mandato in quest'Aula è qualcosa che attiene ad una responsabilità individuale, non è possibile andare oltre un certo limite, non è possibile censurare l'iniziativa individuale di un collega o ritenerla contraria ad un patto di lealtà: essa va considerata per quello che è nel momento nel quale si produce. Vorrei che non esagerassimo, perché altrimenti dalle parole si passa agli atti poiché di atti ve ne sono stati, nei giorni passati, è bene che non si creino i presupposti perché si possano ripetere. *(Applausi Signor Presidente, non volevo intervenire, ma vi sono costretto dalle parole del relatore e in qualche modo faccio seguito a quanto espresso ora dal collega Quagliariello. Mi pare che il relatore abbia una concezione un po' strana dei lavori del Parlamento; sostanzialmente porta avanti questa tesi: siccome in Commissione si sarebbe (dico si sarebbe e poi spiego perché) stipulato una sorta di patto d'onore tra i commissari, l'Aula si deve piegare e non deve discutere gli emendamenti. Intanto faccio mie le considerazioni del senatore Quagliariello, per le quali ogni senatore è evidentemente libero di proporre e di svolgere in Aula tutti gli interventi che vuole. Ricordo al relatore che Ricordo al relatore che l'Assemblea è sovrana. Ricordo inoltre, affinché resti agli atti, che io come Presidente del Gruppo della Lega Nord non ho stretto alcun patto, né d'onore né politico, né di altro tipo, in Commissione.

il senatore Sinisi a dare le giustificazioni di merito per le quali è contrario a determinati emendamenti. Non ho molte speranze che lo faccia, perché vedo che non mi ha ascoltato e quindi probabilmente la volta successiva tirerà fuori ancora la stessa affinché resti agli atti, affermo che non abbiamo stipulato alcun patto, né da uomini d'onore né da gentiluomini, con il senatore Sinisi. Quindi ci riteniamo assolutamente liberi di difendere i nostri emendamenti. *(Applausi dai

fatto che complessivamente questo provvedimento sia condiviso dal Gruppo di Alleanza Nazionale, e mi pare per quello che ho sentito e per il modo con cui si è votato sino ad ora credo anche dagli altri Gruppi, non toglie il diritto ad un senatore che ha presentato un emendamento in Commissione di confrontarsi su questo anche in Aula. Ci mancherebbe altro che togliessimo ai singoli senatori la possibilità di

Complessivamente i Gruppi si sono espressi: l'emendamento non è firmato da tutto il Gruppo, ma da un singolo senatore che aveva il diritto di farlo. Ora andremo al voto e vedremo se l'Aula lo condivide o meno.

Non era sua intenzione - e non lo ha minimamente detto - contestare il diritto di ciascun senatore di presentare un emendamento. Vogliamo soltanto sottolineare che si è svolto su questo argomento nelle Commissioni riunite un ottimo lavoro a cui tutti i Gruppi hanno partecipato e si è trovata una formulazione che in larga misura tiene conto delle posizioni espresse. Le considerazioni svolte dal collega Mantovano nel suo emendamento sono serie.

io vorrei un conforto dal relatore perché, almeno a me personalmente, non risulta chiaro, dal testo proposto, se sia possibile utilizzare i mezzi mediatici per estendere la flagranza e quindi poter arrestare in flagranza di reato chi commette atti di violenza al di fuori degli stadi. Questo emendamento colma tale lacuna. Allora è evidente che, se il relatore mi conferma che non è chiaro che tutto ciò si possa fare anche al di fuori degli stadi, ad esempio nel caso degli episodi di Catania, lo difendo fermamente;

Presidente, ho letto con attenzione la proposta di riformulazione del senatore Castelli, così come ho ascoltato con attenzione le parole che ha pronunciato in precedenza, per il rispetto che gli porto per la funzione che svolge, voglio dirgli che la formulazione che ha previsto è, a mio avviso, specificata nel dettaglio dal decreto-legge in esame, il quale ha esteso non soltanto nello spazio ma anche nel tempo i fatti che consentono l'arresto in flagranza, ancorché differita: si tratta di fatti che accadono 24 ore prima, 24 ore dopo, e anche al di fuori dello stadio, ovviamente con le specificazioni che hanno richiesto

non perché ci sia un patto d'onore ma perché è un buon lavoro, come ha detto il presidente Bianco, che abbiamo fatto insieme e che mi farebbe piacere vedere celebrato in quest'Aula. Mi auguro che le sue preoccupazioni, senatore Castelli, possano essere largamente soddisfatte da queste mie osservazioni. Presidente, ovviamente, visto che il relatore invoca spesso il patto fra gentiluomini, non posso fare altro che fidarmi della sua parola, tenendo presente però una questione: io ritengo che ci sia anche, in questo provvedimento, un *fumus* di incostituzionalità, perché noi riusciamo adesso ad applicare questa fattispecie a chi ha buttato una *molotov* per una squadra sportiva, mentre invece chi la butta in odio agli americani non può essere perseguito sotto questo aspetto. E' la logica di questo Parlamento; ne prendiamo atto.

Degli emendamenti che ho presentato all'articolo 8, di fatto quello che non solo mantengo ma che ha un significato particolare è l'8.8,

un emendamento al quale soprattutto il collega Ciocchetti, responsabile dello sport del mio partito, tiene particolarmente (ed ha ragione). Vorremmo cogliere l'occasione del decreto, che tende a tutelare i cittadini dalla violenza negli e fuori dagli stadi, per tentare di recuperare al massimo la cultura della legalità e dello sport.

una questione che riguarda una specifica squadra). Vorremmo promuovere la cultura dello sport e della legalità da parte delle società sportive. Questo argomento abbiamo il timore che non sia compreso nell'emendamento che la Commissione presenta, testo sembra eccedere nella logica dell'intervento del CONI, delle scuole, dei Ministeri, del Governo. Vorremmo capire se l'Esecutivo, che ha lo stesso obiettivo che abbiamo noi, ritiene che questo tema sia compreso formalmente nel testo nel testo della Commissione o se non sia più opportuno prevedervi espressamente la promozione della cultura della legalità nel calcio anche attraverso convenzioni stipulate da società sportive. È un altro caso nel quale vorremmo, con questo testo, non limitarci alla repressione o alla prevenzione

prevede la non applicazione della sospensione condizionale della pena per quelli che sono stati considerati reati di forte gravità sociale. Riteniamo si dovrebbe evitare

colleghi, l'articolo 8, al comma 1, prevede il divieto per le società sportive di corrispondere, in qualsiasi forma diretta o indiretta, a una serie di soggetti qualsiasi vantaggio, contributo, sovvenzione, facilitazione, eccetera; 4, invece, è prevista una deroga: «In deroga al divieto di cui al comma 1 è consentito alle società sportive stipulare con associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 12 del codice civile (...) contratti

sono magistrati e giuristi certamente illustri - sanno perfettamente che il richiamo all'articolo 12 del codice civile è, a dir poco, inappropriato: se

Vorrei dire che non cambia, perché questa è una formulazione che individua una procedura di identificazione della società che non c'è più. c'è più. Quello che interessa, invece, è la finalità, cioè che le associazioni sportive abbiano tra le finalità statutarie la promozione e la divulgazione dei valori e dei princìpi della cultura sportiva e della non violenza. Quindi, delle due l'una: un invito ai relatori a proporre un emendamento soppressivo; oppure credo sia inevitabile che l'Aula approvi l'emendamento 8.8, proposto dal senatore D'Onofrio e da me.